L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunico che in data 5 maggio 2009 è stato assegnato in sede deliberante alla 7a Commissione permanente, con i pareri delle Commissioni 1a e 5a, il disegno di legge n. 1544, recante «Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019». Le predette Commissioni sono sin d'ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno al fine di procedere all'esame di questo provvedimento. Colleghi, cerchiamo di consentire che i lavori si svolgano in un clima di dignità e che magari si parli tra colleghi in maniera più contenuta.

*(PD)*. Signor Presidente, signori esponenti del Governo, onorevoli colleghi, come in altri interventi del Gruppo Partito Democratico che mi hanno preceduto,

pur in presenza di sezioni dello stesso provvedimento sulle quali abbiamo collaborato, in un confronto significativo che si è svolto all'interno della Commissione anche con risultati...

Prego, senatore Sangalli. Le due critiche principali che mi sento di fare riguardano in primo luogo il fatto che si tratta di un provvedimento che è cresciuto con il passare del tempo, su tematiche tra loro scarsamente legate (talvolta lontanissime), non tenute assieme da una visione strategica economica.

ad affrontare una fase di crisi globale entro la quale si inserisce la specificità strutturale delle difficoltà del sistema Italia. Tale inadeguatezza deriva da sottovalutazioni e da una non perfetta comprensione della crisi che stiamo attraversando, le cui ragioni stanno sì nella finanza globale, ma i cui effetti si manifestano nell'economia reale, soprattutto sulle piccole e piccolissime imprese, quelle imprese - lo voglio dire con chiarezza, perché è stato un tema di confronto nella nostra Commissione - che sono più impegnate sul piano degli investimenti, dell'innovazione e della sfida competitiva. A pagare il prezzo più elevato di questa crisi sono proprio i campioni italiani che sono nella fase di maggiore impegno competitivo ed innovativo. La seconda critica di fondo che mi sento di muovere è che si ha la percezione di un provvedimento complessivamente inadeguato rispetto all'attualità della crisi, ai suoi costi sul piano del capitale umano, del capitale sociale e del capitale imprenditoriale che la crisi ci induce a pagare determinando solchi profondi che si scaveranno soprattutto indebolendo il sistema della piccola e media impresa.

e sui princìpi di natura teorica delle politiche abbiamo cercato di costruire delle situazioni concettualmente nuove (la novità più evidente è rappresentata dalla costruzione della definizione delle reti d'impresa), ma questi principi non si traducono in politiche, non si traducono cioè in quantità, in capacità di investimento o di orientamento degli investimenti da parte dello Stato nei confronti del sistema imprenditoriale italiano. «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese», ed infatti - bisogna riconoscerlo, perché è anche il frutto di un lavoro comune - si produce un significativo passo in avanti sul tema, non solo con la definizione delle reti di imprese argomento che credo avremo modo di votare assieme, già introdotto dal precedente Governo e definito con qualche innovativa chiarezza nella legge n. 33 del 2009 - ma anche con la scelta di intendere le reti, così come i distretti, come forme organizzative finalizzate ad ampliare la competitività dell'intero sistema. lo sforzo compiuto sul piano ordinamentale, ma senza risorse aggiuntive pubbliche un buon obiettivo, come la rete d'impresa - cioè piccole e medie imprese che convergono su obiettivi di competitività rischia di trasformarsi in una organizzazione controllata da imprese più forti che induce altra subalternità strategica e finanziaria. Senza risorse a ciò finalizzate il rischio è che si scriva un buon principio praticandone uno opposto: invece che la collaborazione tra le imprese si pratica cioè la subordinazione tra le imprese. In altre parti di questo provvedimento mi sento di condividere obiettivi e scelte conseguenti. Prendiamo il caso della contraffazione, della sottrazione della proprietà intellettuale, dei reati conseguenti contro chi ha messo in campo inventiva ed investimenti e poi anche contro la fede pubblica che ha acquisito prodotti alterati contro il consumatore finale, inerme e non tutelato. Prendiamo il caso delle affermazioni sul tema della concorrenza nel mercato energetico contenute in questo provvedimento, la cui mancanza è la vera ragione dei costi più alti dell'energia in Italia. In Italia i costi dell'energia maggiori che in altri Paesi non perché non utilizziamo il nucleare, ma perché non abbiamo un sistema competitivo nella gestione e nella distribuzione dell'energia. sono tutti princìpi che condividiamo. Lo stesso dicasi per il tema degli interventi per la reindustrializzazione e il riordino degli incentivi, per alcune linee di tendenza sul commercio internazionale e l'internazionalizzazione delle imprese. Ma se consideriamo il caso dell'energia, per esempio, di cui tanto si parla, ci rendiamo conto che questi obiettivi si affrontano in modo totalmente contraddittorio, nel caso più clamoroso, con ricorso a deleghe al buio al Governo (in questo provvedimento se ne contano almeno otto), con declamazioni ideologiche dai dubbi effetti pratici (è il caso del nucleare), mentre non si interviene sulla sulla libera concorrenza e anzi si procrastinano i termini dell'abuso di posizione dominante del fornitore di energia attraverso il gas, impedendo all'Autorità antitrust di intervenire fin da subito in questo settore. Tuttavia, si annuncia un po' pateticamente che ci lanceremo nell'energia nucleare al di là dell'essere favorevoli o contrari, darà i primi risultati non nella fase in cui abbiamo bisogno di rilanciare il livello di competitività del sistema Paese, ma fra 20-25 anni mentre - aggiungo io - nessun altro Paese che non abbia intenzioni belliche si sta accingendo a costruire nuove centrali nucleari. Sono logiche che contraddicono i principi liberali a cui l'intero provvedimento dice di volersi ispirare. Occorre un mercato trasparente che tuteli il consumatore finale? Si distrugge la *class action* e con un preciso bisturi la si allontana dagli episodi più gravi di truffa finanziaria che hanno coinvolto i consumatori e i risparmiatori nel corso di questi anni (ne sono esclusi, infatti, i casi Parmalat e Cirio). Ci vuole un mercato più competitivo da cui dedurre costi per il consumatore? Si risponde con un regalo alle assicurazioni, con un allungamento *sine die* dell'abuso di dominanza del settore assicurativo, che era stato tolto dalle liberalizzazioni del precedente Governo. Nel settore del gas - lo ricordo ancora - si allungano al 2015 i margini di intervento dell'*Antitrust*, cioè l'impedimento dell'intervento dell'*Antitrust*. in pompa magna che scegliamo il nucleare, adesso che nessun Paese normale ha più fatto tale scelta, i cui effetti saranno apprezzabili fra trent'anni. Nel frattempo, ci teniamo i monopolisti attuali, ben tutelati e senza preoccupazioni di controlli da parte di autorità indipendenti. Se dovessimo vedere questo provvedimento come lo vedrebbe un americano, viene da dire che i titoli li potrebbe aver scritti Obama, ma che i contenuti sono esattamente quelli che avrebbe scritto Bush. È un provvedimento che ha titoli nuovi, buone intenzioni, ma che mal celano vecchie pratiche non trasparenti e non liberali. È un provvedimento ben confezionato, pieno di buone intenzioni, ma anche di numerose dissimulazioni

ma non trovare una sintesi sull'interesse generale del Paese. È un provvedimento che poteva essere una buona occasione per riscrivere le linee di politica industriale; è una buona occasione perduta, con buoni titoli, ma con tante, tante cose che sono diventate deludenti, perché non è stata data al Parlamento la possibilità di lavorarci con serietà e serenità, il che avrebbe reso un Parlamento democratico anche un Parlamento migliorativo dei provvedimenti di politica economica. Debbo purtroppo, tutte le volte che intervengo su argomenti di politica economica, ricordare sempre una grande massima: che la democrazia non è un ostacolo alla buona politica economica, è, come diceva Amartya Sen, l'unica condizione per correggere le politiche economiche sbagliate. Siccome nessuno ha il dono della verità, sopratutto nella politica economica se più pareri si confrontano talvolta si riescono anche a migliorare le politiche economiche sbagliate.

il provvedimento in discussione, nonostante la crisi finanziaria che è stata comunque affrontata con prontezza e responsabilità dal Governo Berlusconi, offre risposte concrete sulla questione dello sviluppo economico. È, infatti, importante sottolineare come il Governo abbia con lungimiranza presentato il provvedimento in esame in una manovra economica varata prima dell'estate e che, in buona parte, ha avuto già attuazione; dunque, prima che gli effetti della crisi fossero tangibili a tutti. Questo provvedimento realizza una forte valorizzazione delle specificità del nostro Paese che, allo stesso tempo, costituiscono il motore del nostro sistema produttivo. È evidente come le disposizioni in esso previste affrontino in maniera riformatrice tematiche che attendevano da tempo maggiore attenzione. In particolare, si pone rimedio all'inefficacia sinora dimostrata dalla legislazione in materia di lotta alla contraffazione. È previsto un rafforzamento dei sistemi produttivi e delle reti d'impresa, s'introduce una maggior tutela del diritto di proprietà intellettuale, viene riformata la disciplina degli incentivi e si introducono misure di sostegno al commercio internazionale e al processo di internazionalizzazione delle imprese. È di tutta rilevanza la previsione della delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti d'impresa, con l'obiettivo di semplificare la normativa ed agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. È infatti essenziale accompagnare lo sviluppo del sistema produttivo con una indispensabile semplificazione delle norme. In merito alle altre misure previste nel testo, voglio qui sottolineare come, facendo riferimento all'internazionalizzazione delle nostre imprese, sia stato inserito opportunamente un graduale riordino dei tanti enti ed organismi, affinché gli stessi possano essere davvero funzionali allo sviluppo del commercio estero e non si pongano invece quali intermediari di comodo, con la sola finalità di mantenersi in vita e dunque di tenere in piedi un apparato burocratico costoso che non produce servizi alle imprese. Altro elemento di indiscutibile importanza è l'inasprimento delle sanzioni per reati da contraffazione, reati che non solo ledono l'immagine delle nostre aziende, ma in moltissimi casi costituiscono un pericolo o producono danni alla salute, poiché le merci contraffatte vengono realizzate senza alcun rispetto della salute pubblica. Di certo, queste misure daranno maggiore fiducia alle nostre aziende, che in questo momento, oltre a dover subire le conseguenze della crisi finanziaria, devono quotidianamente confrontarsi su un mercato globale dove operano anche aziende cosiddette fantasma, senza regole né norme precise da rispettare, mentre le nostre imprese, che producono qualità ed eccellenza dal tessile all'agroalimentare, a tanti altri settori, vedono la loro azione stretta da un legislazione europea che sa porre paletti al proprio interno, ma non sa affrontare con la stessa tenacia la competizione scorretta di alcuni Paesi extracomunitari. L'organicità del provvedimento in questione si palesa in modo incisivo nel momento in cui dispone misure nei confronti del sistema energetico, sistema che ha sempre denotato una scarsa capacità di rinnovamento, nonostante gli esempi dei vicini Paesi dell'Unione europea che hanno, grazie all'energia nucleare per usi civili, sostenuto lo sviluppo e il loro mondo produttivo. Nel testo è presente, infatti, la delega al Governo per il ritorno del nucleare in Italia, ritorno che non era più plausibile prorogare nel tempo di fronte ad un *gap* energetico che ci ha resi poco competitivi, nonostante le nostre aziende energetiche possano collaborare a pieno titolo a progetti inerenti il nucleare da realizzarsi all'estero. Non è più accettabile che un Paese industrializzato come il nostro debba dipendere per gran parte del suo fabbisogno energetico da Paesi quali la Russia e l'Algeria. Ciò comporta che i costi energetici in Italia siano per almeno il 20 per cento maggiori rispetto al resto d'Europa. Ciò colloca le nostre aziende in una posizione di svantaggio rispetto al sistema produttivo di altri Paesi e concede meno *chance* di competitività ai nostri prodotti sui mercati esteri. Per troppo tempo, cari colleghi, siamo stati ostaggio di una politica ambientale del tutto ideologica e contraria *a priori* allo sviluppo del Paese. Una politica ambientale che ha individuato da sempre nell'applicazione del nucleare una possibile catastrofe, per poi non accorgersi o far finta di nulla rispetto ai gravi danni procurati da un inquinamento che in casa propria vedeva la presenza di una miriade di discariche abusive e rifiuti ammassati nelle strade, con la criminalità organizzata a gestire il malaffare. I cosiddetti ambientalisti ed i loro rappresentanti politici, che in passato hanno avuto anche incarichi di Governo, ci mostravano i loro telefoni cellulari alimentati con energia solare e non vedevano la spazzatura ammassata, che rappresentava un pericolo costante per la salute di migliaia di persone. Anche in questo caso, il Governo Berlusconi ha risposto con tempestività ed incisività, chiudendo la brutta pagina dell'emergenza rifiuti in Campania. È giunto, però, il momento di affrontare il tema dell'energia ed il provvedimento in esame legifera, introducendo regole certe ed avendo grande rispetto ed attenzione per l'ambiente, l'ambiente, nella consapevolezza che il nostro patrimonio paesaggistico, culturale, storico ed architettonico è e rimane intoccabile. Allo stesso tempo, il disegno di legge in esame dispone norme volte ad innovare un sistema da troppo tempo ingessato, che non ci ha permesso sino ad ora di guardare al futuro e dedicarci a quelle forme di energia, come il nucleare e le energie rinnovabili, che possono costituire quel binomio energetico che favorisce lo sviluppo e può contribuire sia alla difesa dell'ambiente, che a far diminuire il costo dell'energia elettrica. Tutto ciò sarà garantito, cari colleghi, da un Governo che ha saputo dimostrare ampiamente le sue capacità e che saprà, anche in questo caso, dare una soluzione definitiva all'annoso e non più rinviabile problema dell'approvvigionamento delle fonti energetiche.

rappresentanti del Governo, stiamo parlando di un provvedimento che ha animato il dibattito in Commissione ed anche all'interno delle realtà produttive di questo Paese,

che il disegno di legge riguarda disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

hanno come obiettivo solo e soltanto lo sviluppo delle imprese. Quando vengono inserite all'interno di un disegno di legge norme relative al settore ferroviario, riteniamo che quel settore - oggi in fase di grande espansione sul mercato nazionale ed internazionale

e altri ancora. Vi è soprattutto a livello nazionale l'esigenza di armonizzare alcune realtà in un mercato mondiale profondamente cambiato che sta creando grossi problemi alle imprese italiane.

Stato, importano in questo Paese, spesso e volentieri anche con riflessi di carattere criminoso, prodotti che vanno ad incidere negativamente sullo sviluppo delle nostre imprese.

di un articolato che vada incontro anche alle esigenze poste giustamente dall'opposizione affinché si giunga ad una condivisione nella formulazione degli stessi articoli. Ho sentito da più parti in questi ultimi anni e mesi la denuncia che viene dal nostro Paese e dalle categorie che hanno portato recentemente il tema dell'energia ad un dibattito a livello internazionale.

nazionale e delle piccole e medie imprese italiane, che si sono conquistate spazi a livello mondiale ed internazionale e che vanno oggi sostenute e difese nel processo di riconoscimento a livello europeo. Qualche Paese sta facendo operazioni di sostegno esclusivo delle produzioni nazionali: noi abbiamo sempre tenuto conto dei processi

di votazione degli emendamenti e degli articoli si tenga conto che con il disegno di legge in esame compiamo un passo significativo. Voltiamo pagina, rimettiamo l'Italia, come giustamente deve essere non solo a livello nazionale ma anche internazionale, nel novero dei Paesi più

nel quadro della manovra di finanza pubblica per l'anno 2009 e per il triennio successivo. È un provvedimento che sin dall'inizio ha affrontato

con elementi innovativi anche per quanto riguarda l'agevolazione alla reindustrializzazione di aree in crisi, e certamente anche il tema significativo in questo quadro del riordino degli incentivi. Questa è la prima parte significativa di un provvedimento che quindi riforma, se vogliamo in maniera strutturale, il sistema dell'industrializzazione e degli incentivi nel nostro Paese. La seconda area - veniva sottolineato anche prima dal presidente Cursi - è quella che riguarda il commercio internazionale e l'internazionalizzazione delle imprese, tanto più significativa oggi alla luce della crisi mondiale, che è sopratutto una crisi dei nostri principali *partner* internazionali, alla quale le imprese italiane stanno rispondendo meglio delle imprese di altri Paesi occidentali. Valgano per tutti due esempi che credo significativi e che ci devono confortare sulla tenuta del nostro sistema industriale e sulla capacità di reazione dello stesso anche ai nuovi contesti globali.

quando la stessa stava per essere annessa da una grande casa automobilistica americana. Ebbene, oggi si sta verificando esattamente il contrario: è la FIAT che va in salvataggio della Chrysler, forse dell'Opel, probabilmente di altri rami della General Motors in Sud America. Questo ci fa capire come le imprese italiane siano in condizione di reagire. Il secondo esempio che voglio portare all'attenzione di quest'Assemblea riguarda proprio il dinamismo delle nostre imprese all'estero; ai primi di aprile, nel momento più acuto della crisi internazionale, circa 1.000 imprenditori italiani sono andati in missione di sistema a Mosca e tante altre missioni si fanno ovunque nel mondo. Questo dimostra come il nostro sistema industriale può e sa reagire alla crisi globale e va aiutato in tal senso. In questa area del commercio internazionale e della internazionalizzazione delle imprese sono comprese anche alcune deleghe estremamente significative per il riordino degli enti, degli incentivi e per quanto riguarda il Testo unico sul commercio con l'estero e la tutela del*made in Italy*, anche attraverso un'opera più efficace di lotta alla contraffazione e di difesa dei marchi. Questa è la terza area del provvedimento, che reputiamo molto significativa e su cui i colleghi si sono soffermati. La quarta area investe lo sviluppo energetico del Paese, sia per quanto riguarda lo sviluppo dell'energia rinnovabile sia per quanto concerne il ritorno all'uso dell'energia nucleare del nostro Paese. Il provvedimento presentato, come ho detto, il 2 luglio e poi scorporato, stralciato come provvedimento autonomo, è in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, ormai -

poi al Senato, in Commissione e oggi in Aula, è intervenuto in maniera efficace. Se i colleghi dell'opposizione vedono il testo iniziale presentato dal Governo, si renderanno conto essi stessi di quanto lavoro è stato svolto, prima alla Camera e poi in Commissione

che considera centrale per lo sviluppo del Paese, si è posto con un atteggiamento positivo, costruttivo, aperto al dialogo nei confronti del Parlamento, di tutti i Gruppi e di tutti i parlamentari. Per questo il provvedimento è via via cresciuto

intendo soffermarmi in conclusione. Il provvedimento riguarda certamente l'utilizzo dell'energia nucleare nel nostro Paese, ma soprattutto l'uso di ogni forma energetica, e si sofferma con attenzione sul *mix* energetico che l'Italia deve raggiungere nei prossimi anni; un *mix* che ci permetta di rispettare meglio l'ambiente, di ridurre le emissioni di anidride carbonica in sintonia con gli

l'utilizzo e la produzione di energia rinnovabile nel nostro Paese fino a raggiungere un *mix* energetico che possa equilibrare la bolletta elettrica italiana, anche per quanto riguarda la bilancia commerciale: un *mix* energetico formato dal 25 per cento di energia rinnovabile e dal 25 per cento di energia nucleare. Il nostro Paese e le nostre imprese sono in condizione di farlo, come dimostra anche il percorso che una grande impresa elettrica come l'ENEL ha fatto in questi anni, internazionalizzandosi e diventando un grande gestore di di energia nucleare all'estero (in Spagna, Slovacchia, verosimilmente anche in Francia e in Bulgaria): e questo dimostra che lo si può fare in Europa, e quindi anche in Italia. Penso che su questa strada possiamo incamminarci.

si appresta a valutare gli emendamenti che saranno sottoposti a questa Assemblea, nella certezza che alla fine il lavoro sarà migliore e che ciò possa contribuire affinché l'impresa italiana e il nostro Paese confrontarsi al meglio in un contesto difficile. Il provvedimento è stato presentato il 2 luglio, prima che si verificassero i più gravi eventi e le più pesanti conseguenze della crisi economica ed anche per questo è stato migliorato nel corso degli ultimi mesi. era allora ed è ancor più oggi un provvedimento assolutamente necessario, che può consentire alle nostre imprese di reagire meglio alla crisi dei consumi mondiali e, forse, di cogliere meglio di altre imprese e di altri Paesi le nuove opportunità che ci saranno. Forniamo loro un contesto legislativo più adeguato, perché esse - che sono gli attori dell'economia - possano utilizzarlo al meglio. sottolineo il mio ringraziamento ai senatori della Commissione industria del Senato per il lavoro che abbiamo svolto in questi mesi, che ritengo proficuo per il bene del Paese. Con questo atteggiamento costruttivo,

conferma dell'importanza strategica di questo provvedimento, che ha avuto un *iter* complesso in Commissione, con un susseguirsi di emendamenti e subemendamenti, il cui esito si è potuto però concludere soltanto stamattina: solo alle ore 9 di questa mattina, infatti, è stato disponibile il fascicolo degli emendamenti. A ciò dobbiamo aggiungere

mi induce a chiederle, a nome del Partito Democratico, che l'esame degli emendamenti e le successive votazioni possano aver luogo a partire dall'inizio della seduta di oggi pomeriggio. Il Gruppo del Partito Democratico, infatti, non è assolutamente in grado di esprimere un'opinione meditata

il disegno di legge al nostro esame risulta dall'unificazione di due proposte di legge di iniziativa parlamentare ed è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati il 29 aprile scorso. Esso dispone un'estensione del diritto di voto a domicilio degli elettori impossibilitati a spostarsi autonomamente dalla propria dimora. La normativa vigente in materia assicura l'esercizio di tale diritto

In sostanza, il requisito della necessaria dipendenza da apparecchiature elettromedicali non ha consentito di comprendere tra gli aventi diritto al voto a domicilio una fascia consistente di cittadini non in grado, comunque, di recarsi al seggio elettorale né in modo autonomo, né con l'aiuto dei supporti messi dei supporti messi a disposizione dai Comuni italiani: si tratta dei cosiddetti disabili intrasportabili che, per le loro gravissime condizioni di salute che li costringono alla immobilità, non possono spostarsi fuori dalla propria dimora.

Questo provvedimento è una legge che attua l'articolo 48 della nostra Costituzione, che al secondo comma recita: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.». E dove c'è un dovere civico deve corrispondere un dovere dello Stato e delle istituzioni di mettere tutti i cittadini nella condizione di poter esercitare questo loro dovere civico. la stessa Costituzione, al quarto comma dell'articolo 48, afferma che il diritto di voto non può essere limitato. Quindi, rendere possibile agli intrasportabili il diritto di voto è davvero

forse anche per farci perdonare del tempo che abbiamo lasciato trascorrere in Parlamento senza occuparci di una questione tanto importante. L'articolo 1 modifica il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1. Alla lettera *a)*, attraverso una modifica del comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge, si intende dare maggiore compiutezza al dettato costituzionale, estendendo la platea dei soggetti titolari del diritto di voto a domicilio agli elettori affetti da gravi patologie che si trovino, presso la propria dimora, nella duplice condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche. Potranno quindi votare al proprio domicilio anche gli elettori affetti da infermità tali da rendere impossibile l'allontanamento dalla propria abitazione o che comunque comportino il rischio di aggravamento dello stato fisico. Alla lettera *b)*, che modifica il comma 3 del citato decreto-legge, si interviene sulle modalità di presentazione della richiesta di ammissione al voto domiciliare. Si prevede infatti che l'elettore il quale intende esprimere il proprio voto presso l'abitazione in cui dimora

nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione in carta libera nella quale si indicano il motivo per cui richiede il voto domiciliare e l'indirizzo presso il quale intende esercitare il diritto di voto, nonché un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, per l'accertamento delle situazioni di infermità con prognosi di almeno sessanta giorni, decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature. Tale disposizione origina dalla volontà, sottolineata in particolare dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, di contenere la platea dei soggetti destinatari, assicurandosi, con apposito giudizio medico, l'effettiva intrasportabilità dell'infermo. La lettera *c)* introduce un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 1 del decreto-legge n. 1 del 2006. Esso dispone misure sanzionatorie nei confronti di false dichiarazioni da parte del funzionario medico, con la sospensione del rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi. Di rilievo è anche la modifica apportata alla lettera *e)*, che introduce un nuovo comma 9-*bis*, sempre all'articolo 1 del decreto-legge. Si dispone che la commissione elettorale circondariale può disporre che il voto dei soggetti che hanno esercitato il loro diritto al voto presso la propria dimora venga raccolto dal seggio speciale che opera negli ospedali o case di cura ubicate nelle vicinanze delle abitazioni di tali elettori. Il disegno di legge è stato approvato in Commissione affari costituzionali nella seduta di ieri con il voto unanime di tutti i suoi componenti. Auspico pertanto una rapida approvazione del provvedimento, che consenta l'entrata in vigore della disciplina in tempo utile perché possa trovare applicazione fin dalle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

ad adottare ogni misura necessaria, anche attraverso opportune campagne di informazione, al fine di rendere per quanto possibile operativo, in via sperimentale, l'esercizio del voto domiciliare per gli elettori ammessi, già a partire dalla prossima tornata elettorale fissata per i giorni 6 e 7 giugno del corrente anno, nonché ad assicurare in ogni caso una piena attuazione della legge per le successive elezioni.

un'elevata frequenza, trattamenti ad alto contenuto tecnologico), per cui non può abbandonare il domicilio.

che si registra in svariate parti del Paese - per molti di questi malati l'insieme di queste terapie può svolgersi a casa,

avremmo potuto votarlo almeno 15 giorni fa. Oggi siamo al limite per poter permettere l'esercizio di voto a questi nostri concittadini già dalla prossima scadenza elettorale.

se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge; però, in realtà, l'esercizio del voto è per alcuni cittadini molto difficile. Ci tengo a lasciare agli atti una lettera che fu inviata a dicembre al Presidente del Consiglio. Chi la firma è Severino Mingroni. Si definisce così: «Sono un disabile gravissimo ed ho tante di quelle gravi invalidità - ho la LIS (*Locked-in Syndrome*) da trombosi alla arteria basilare, dalla fine quasi dell'ottobre 1995 - il che comporta che l'andare a votare al seggio elettorale è una vera e propria tortura fisica e psicologica. Caro signor Presidente del Consiglio, vorrei provare a documentarle con un video una tale tortura fisica "democratica", pure perché, in questo modo, avrà forse una chiara idea del grave "stress" psicologico a cui siamo sottoposti io e i miei familiari quel giorno. Essendo io un abruzzese residente a Casoli in provincia di Chieti, mi è sembrato opportuno votare al seggio per le elezioni regionali del 14 e 15 dicembre 2008. Di questa mia tortura "democratica" farò fare un video - probabilmente dai miei amici radicali - e glielo manderò. Da quando ho la LIS, sono andato a votare solo nel giugno 2005, per il *referendum* sulla legge 40, ed è tutto documentato su Internet da un servizio fotografico nel mio sito: nonostante ci fosse un bel sole e facesse caldo, fu, per me e la mia famiglia, un vero calvario. Infatti, anche se il mio seggio dista poco dalla casa del sottoscritto, Casoli non è un paese in pianura; quindi, devo pure farmi trasportare da una auto apposita per espletare un semplice ed elementare mio diritto; e poi, mi auguro proprio che, il giorno del voto dello scrivente, non nevichi o piova forte o faccia molto freddo, affinché la tortura "democratica" sia meno tortura. Votare a domicilio perciò sarebbe per me una ottima opportunità che mi eviterebbe un notevole stress psicofisico; tenga pure conto che, da quando sto qui al computer, mi sento una persona normale come lei, caro signor Presidente del Consiglio, mentre, quando vado a votare al seggio, mi sento solo un disabile gravissimo, anche tetraplegico e muto».

la legge a prima firma dell'onorevole Rita Bernardini (radicale nel Gruppo PD), poi sottoscritta da parlamentari di tutti gli schieramenti, fosse approvata e quindi valida per le elezioni di giugno. Ci fu la risposta del Presidente del Consiglio: c'è stata infatti la risposta del Governo che ha fatto sì che questa legge venisse approvata, anche se nei tempi limite che abbiamo appena detto. La risposta è oggi anche di questo Parlamento, che fa onore a se stesso e, per un volta, ci vede uniti ad approvare una legge per i cittadini.

non soltanto per la passione con cui in Commissione ha affrontato la questione, ma anche per quanto ha detto poco fa, cioè che questa tutto è tranne che una leggina. Anzi, si potrebbe dire che è il recupero di un diritto civile negato per sessant'anni a migliaia di cittadini italiani. Sicuramente una volta non c'erano tutte le tecnologie necessarie affinché anche chi ha problemi fisici potesse godere appieno di quella che viene chiamata oggi una vita indipendente, che include anche il godimento dei diritti di elettore.

proposti da Alleanza Nazionale non raggiunsero il *quorum* per poche migliaia di voti. In quello stesso anno i radicali denunciarono la presenza nelle liste elettorali di milioni di italiani morti

Dunque, chi non era più sul suolo patrio e, se ci si crede, anche detentore di anima, in questa Repubblica ha condizionato una tornata elettorale, mentre allo stesso tempo migliaia di italiani, pienamente capaci di intendere e di volere, come

Due settimane fa i radicali hanno pubblicato un libro, intitolato «La peste italiana», che proprio di questo parla: mette in sequenza sessant'anni di progressiva occupazione delle istituzioni pubbliche da parte dei partiti politici volti esclusivamente a mantenere se stessi al potere e a non dare la possibilità ai cittadini italiani di godere dei propri diritti,

che hanno fatto della loro individualità non qualcosa da far strumentalizzare politicamente, ma una militanza politica quotidiana per il rispetto della Costituzione e non per l'allargamento dei diritti di chi vive in condizioni difficili, ma per il pieno godimento dei diritti in quanto individui. L'Italia all'inizio dell'anno ha ratificato la Convenzione

e anche, in certi casi, psichiche complesse. Questa legge recupera il maltolto di sessant'anni di partitocrazia. Speriamo di raggiungere presto questo obiettivo, ma saranno le istituzioni, come chiede l'ordine del giorno che abbiamo adottato ieri all'unanimità,

all'imminente applicazione della norma, pur nella ristrettezza dei tempi, in una forma concretamente e pienamente esecutiva, seppur seppur sperimentale nella parte che riguarda gli elettori non dipendenti da apparecchiature elettromedicali, ma affetti da gravissime infermità tali da non permetterne l'allontanamento da casa, sempre nella piena realizzazione di quanto disposto dalla volontà del Parlamento e in attuazione di quei princìpi democratici e costituzionali ricordati anche questa mattina in Aula. Procederemo fin da subito anche nello spirito e nei contenuti dell'ordine del giorno G100, che accogliamo e facciamo nostro. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo

intervengo soltanto per confermare a nome mio e del mio Gruppo un voto favorevole nei confronti di una legge che giudichiamo di civiltà; qualsiasi disabile è comunque una persona e, come tale, ha i diritti di tutte le altre persone. Ringrazio il relatore e tutti quelli che si sono occupati di tale provvedimento. Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, il Gruppo dell'Italia dei Valori vota con convinzione questo provvedimento che ricostruisce, dopo una sessantina d'anni, un diritto costituzionale sancito dell'articolo 48, su cui già molti colleghi si sono espressi. Vorrei fare una sola osservazione: è estremamente positivo che sia restaurato il diritto di voto per migliaia e migliaia di persone che non ne hanno goduto per motivi di varia natura. La scelta è stridente, nel senso che contrasta con la prassi passata del Parlamento, che ha prodotto una legge elettorale che vanifica il diritto di voto. Quindi, è simpatico avere il diritto di voto; è meno simpatico scoprire che questo diritto di voto è vanificato tanto che milioni di cittadini sono stati privati della loro legittima rappresentanza politica.

Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico voteranno convintamente a favore del disegno di legge che stiamo esaminando. Non c'è bisogno di di aggiungere molte parole. Si tratta, con questo disegno di legge, di eliminare una piccola grande ingiustizia: una piccola ingiustizia, perché riguarda alcune migliaia di cittadini; una grande ingiustizia perché, grazie alla disattenzione che si è avuta nei confronti di questo aspetto, per molti anni persone che spesso si trovano già private delle libertà fondamentali di potersi muovere e vivere una vita normale si sono trovate anche ingiustificatamente ed ingiustamente private di un diritto politico essenziale, che è quello di partecipare alle operazioni di voto. Il disegno di legge risolve la questione. Probabilmente grazie all'ordine del giorno G100 e G100 e ad un atteggiamento di collaborazione che vi è stato in Commissione tra la maggioranza, l'opposizione e anche, onestamente, il Governo (a tale riguardo ringrazio il Sottosegretario), sarà forse possibile già da subito, con una efficace azione di comunicazione, riuscire ad intervenire.

Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà. Mi rifaccio a quanto detto dal relatore, presidente Vizzini, sull'importanza di questa legge, che perfeziona il diritto di voto per alcuni cittadini che si trovano in situazioni particolari. Vorrei sottolineare che in questo campo l'Italia è sicuramente tra i Paesi del mondo che hanno un procedimento elettorale maggiormente

urne è merito dei cittadini italiani, che sentono l'impegno di votare nelle varie tipologie di elezione, ma è anche merito di un sistema che è stato elaborato nel corso degli anni e che questa legge rende ulteriormente garante dei diritti dei cittadini. Vorrei ricordare che l'Italia è, appunto, molto in alto nella classifica dell'affluenza alle urne:

Per queste ragioni, il Popolo della Libertà voterà convintamente a favore

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo reso alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:"; che all'articolo 3, comma 2, lettera *i)*, dopo le parole: "di risorse", siano aggiunte le altre: "che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità"; che all'articolo 3, all'alinea del comma 2, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" vengano aggiunte le altre: "salvo quanto previsto dal comma 2-*bis*" e che sia inserito il seguente comma: "2-*bis*. L'attuazione del criterio di cui alla lettera *l)* del comma 1 è condizionato al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria"; che all'articolo 4-*bis*, comma 13, vengano soppresse le seguenti parole: "nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate"; che all'articolo 14, comma 2, lettera *q)*, dopo la parola: "previsione" siano inserite le seguenti: "nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo"; - che all'articolo 16, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici spa e dell'Acquirente Unico spa da parte dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."; che all'articolo 16, comma 14, lettera *c)*, l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: "Ai componenti del comitato interistituzionale non spetta alcun compenso né rimborso spese comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; - che all'articolo 16 il comma 23 sia sostituito dal seguente: "Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 nonché l'avvio e il monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di tre milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica."; che all'articolo 17, comma 3, siano soppresse le parole: "è indipendente" e venga aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1, senza nuovi e maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui al comma 15."; - che all'articolo 18, comma 17, dopo le parole: "non costituiscano oneri specifici a carico dei consumatori" siano inserite le altre: "né direttamente né indirettamente."; che all'articolo 20, al comma 4, le parole: "nonché degli oneri di cui all'articolo 17, comma 9" vengano soppresse; - che all'articolo 27 venga sostituito l'ultimo periodo con il seguente: "All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica."; - che all'articolo 27-*bis*, comma 1, il secondo periodo venga soppresso e il terzo periodo venga sostituito dai seguenti: "Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2". La Commissione esprime poi parere di contrarietà semplice sugli articoli 16, comma 1 l-*bis*, 18-*sexies* e 33-*decies*. La Commissione osserva che il rinvio alla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2008, contenuto nel comma 16 dell'articolo 17, andrebbe aggiornato con i riferimenti all'ultima legge finanziaria per l'anno 2009».

di materiale rotabile presenti su vasta parte del territorio nazionale, a seguito di talune iniziative assunte da parte di Trenitalia spa L'interrogazione è rivolta ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze,

due barconi con 150 persone a bordo hanno lanciato la richiesta di soccorso in acque internazionali, uno a 56, l'altro a 45 miglia a sud

giusto moralmente, oltre che politicamente, che, anche in questi momenti, dal Senato e dalla sua Presidenza - che sollecito in questo senso - venga un segnale al Governo italiano per un intervento tempestivo, affinché in primo luogo siano garantite la sicurezza e la salvezza delle persone coinvolte.